ed è stato per tre legislature senatore in quest'Assemblea. Sottosegretario di Stato per l'industria, poi agli affari esteri in due successivi Governi, è stata una personalità, come hanno evidenziato anche i suoi oppositori politici dell'epoca, che ha onorato la città di Firenze e le istituzioni

abbiamo notato un attacco feroce ad un Paese, l'Azerbaigian, con il quale abbiamo stretto importanti rapporti commerciali, nonché energetici, che mettono il nostro Paese al riparo da ogni tipo di rischio

nelle affermazioni, erronee riprese di risoluzioni internazionali. Le risoluzioni ONU in merito al conflitto azero-armeno dicono l'esatto opposto di ciò che in quella trasmissione è stato sostenuto. Noi crediamo che non si possa fare informazione in questo modo; che non si possano fare interviste a membri di questo Parlamento e poi tagliuzzarle ed incollarle in modo che il senso finale sia addirittura distorto. Se si vuole fermare una importante opera, che garantisce l'indipendenza energetica del nostro Paese, lo si faccia politicamente in quest'Assemblea, ma non con una informazione distorta, addirittura sulla televisione di Stato. Essendo anche Presidente del Gruppo interparlamentare di amicizia

sospendo la seduta fino alle ore 18. *(La seduta, sospesa

per l'impegno profuso a far sì che i tempi di disamina del provvedimento fossero i più veloci possibili, nel rispetto della necessità - imponderabile per tutti - di rispondere con concretezza alle esigenze urgenti e di prospettiva delle comunità delle Regioni così duramente colpite dal susseguirsi di quei drammatici e violenti terremoti. Abbiamo dovuto collegare due gravissimi eventi sismici, distanziati nel tempo e con caratteristiche diverse, tanto che il Governo - che ringrazio per il supporto al lavoro della Commissione - si è visto costretto ad emanare due distinti decreti-legge, che abbiamo ricondotto a sintesi con il provvedimento che ora stiamo affrontando. Non posso non segnalare, quindi, il clima positivo a cui hanno contribuito tutte le forze politiche presenti nella Commissione bilancio,

colpiti dal dramma di quelle popolazioni. È un clima positivo che ha portato a un dibattito condiviso e all'approvazione di circa 25 emendamenti a un testo già molto completo. Pregherei l'Assemblea di abbassare la voce perché è difficile seguire la presentazione di questo disegno di legge. Prego, senatore.

che tutte le norme previste dal Governo potessero essere migliorate e rese subito operative dalla conversione in legge di questo decreto-legge. Il primo decreto-legge, che ha provato a dare struttura all'emergenza e alla ricostruzione,

Il secondo decreto-legge ha completato gli interventi del primo, prendendo atto di un secondo terremoto che ha esteso in maniera straordinaria, purtroppo, il territorio colpito da entrambi i sismi.

e oggi sottoposte anche a una condizione climatica delicata e difficile, stando in montagna. Il primo decreto-legge è stato considerato da tutti molto positivo.

alle tante questioni che un terremoto come quello poneva; tante questioni che, purtroppo, l'esperienza dei precedenti terremoti ha visto accumularsi attraverso numerose e successive sovrapposizioni legislative e che invece in quel decreto-legge venivano immediatamente prese in considerazione. il secondo decreto-legge si sono raccolti anche elementi di dibattito di quei primi giorni, intervenendo già sulle popolazioni colpite dal primo terremoto, tenendo conto che in quel territorio la "fabbrica", quella che deve ripartire per prima, è il sistema agroalimentare, il sistema dei parchi, il sistema ambientale. È il sistema produttivo legato alla terra e all'ambiente quello che deve ripartire immediatamente. Sono stati pertanto previsti immediati interventi per assistere i lavoratori che operano nelle campagne, dando loro la possibilità di non lasciare le produzioni, ma di ripartire subito, di non lasciare neanche per un attimo le risorse a risorse a loro disposizione e sulle quali lavoravano. Analogamente, con il secondo decreto-legge si è intervenuto immediatamente per consentire che il sistema scolastico fosse un elemento di coesione e potesse ripartire senza dividere le comunità, con quella eccezionalità necessaria quando

l'idea di interventi integrati, di interventi che garantiscano la sicurezza (la terza parola d'ordine) nella trasparenza (la quarta parola d'ordine) e nella legalità (la quinta parola d'ordine). L'idea è che questo decreto-legge, questo intervento che proponiamo all'Assemblea

ne sono due che costruiscono questo decreto-legge. Una è la scommessa di ripetere la buona ricostruzione fatta in Emilia-Romagna: un esempio positivo, un esempio che ha tenuto conto dell'idea che, per mantenere le comunità, si debba partire dal metterle nelle condizioni che il tessuto economico e sociale sopravviva al trauma del terremoto e possa ripartire immediatamente l'economia, che trattiene le popolazioni. La seconda buona prassi, considerata esemplare per questo decreto-legge, è la sorveglianza degli appalti necessari per la ricostruzione, che sono mutuati dall'esperienza Expo. queste due coordinate, l'esperienza positiva del terremoto in Emilia-Romagna e l'esperienza positiva di Expo, sono le coordinate sulle quali si basa questo decreto-legge, che tenta di dare una risposta integrata ed organica alla ricostruzione. Ma c'è un elemento di fondo che prova a dare un'ispirazione, uno spirito, una coscienza a questa ricostruzione. L'idea è che territori, già duramente colpiti e fragili sul piano demografico,

Per questi territori, che già soffrono di una debolezza e di una fragilità demografica, è tanto importante quanto necessario agire con velocità, costantemente e contemporaneamente su tutti i versanti

all'interno di questa iniziativa legislativa c'è anche questa attenzione, questo spirito di fondo: provare a rallentare, a trattenere, a invertire il processo di impoverimento demografico, che è già in atto in quei territori.

Si sentono simili a quei territori del Mediterraneo che, dopo le rivoluzioni democratiche, sono diventati purtroppo Paesi da cui stare lontani. Hanno addirittura questa paura

che lì bisogna aiutare contribuendo all'economia locale, essendo presenti, tornando ad essere presenti, anche solo come turisti. È un grido di allarme, perché la paura della popolazione a ritornare in quei luoghi (quelli che lì non abitano, che non sono abituati a convivere con una terra che trema) che trema) è difficile da superare e si supera con l'esempio. Ci hanno chiesto questo. Ci hanno chiesto: ricostruite, ma ricostruite anche moralmente, ricostruite con la vostra presenza, ricostruite con la vostra partecipazione l'immagine, l'idea, la vocazione di questi territori. nostro esame si sforza di mettere al primo posto il mantenimento dell'integrità di questo tessuto umano e civile perché soltanto se si mantiene tale integrità, se si mantiene questa speranza, si può restituire forza al tessuto sociale ed economico. Per la prima volta, con questo decreto-legge, si interviene dopo un terremoto consentendo non solo la ricostruzione di tutte le prime case ma anche,

integro il tessuto sociale delle istituzioni del territorio. Molti degli interventi sono finalizzati a consentire che i sindaci, che sono i soggetti ai quali le popolazioni si rivolgono, i più vicini rappresentanti dello Stato, non siano inermi e possano agire, possano essere sostenuti sia con l'integrazione di personale tecnico-amministrativo a loro supporto

si sono spostati, per dare loro la speranza che potranno rientrare rapidamente a vivere e a produrre nelle loro comunità. La tenuta dei sindaci, per noi, per la Commissione che ci ha lavorato e ragionato, è un elemento fondamentale perché a partire da quel tessuto istituzionale locale si costruisce la tenuta del tessuto umano come contributo ulteriore. Poi, per quanto abbiamo previsto, come ho detto all'inizio, una particolare attenzione per il settore agricolo. È intervenuto rapidamente il ministro Martina su questo tema e la Commissione ci ha lavorato ulteriormente anche allargando i settori, ad esempio con un emendamento che è stato approvato questa mattina sul settore equino equino che era stato escluso temporaneamente. Tale emendamento, presentato da una forza di minoranza di questo Parlamento, è stato considerato importante. Il tessuto economico, non solo per la parte agricola e agroalimentare, è tenuto presente e per questo vi è una forte attenzione a consentire delocalizzazioni temporanee di ogni struttura commerciale, purché all'interno dello stesso Comune.

Sosteniamo quindi, nell'emergenza, tutti i lavoratori delle imprese. Stamattina abbiamo esteso ai lavoratori dipendenti da ogni soggetto, non solo dalle imprese, tutte le provvidenze previste.

le piccole imprese già esistenti o a strutturare meglio e salvare quelle grandi, ma anche a rendere quel tessuto economico attrattivo, grazie a strumenti che la legislazione nazionale, recentemente aggiornata, ha messo a disposizione delle aree di crisi. Sarà possibile istituire in quei territori le aree di crisi complessa che abbiamo previsto già per le aree industriali in tutto il territorio nazionale, aree che si sono indebolite perché è cambiata la vocazione industriale. Non è un elemento da poco, è un elemento che dà l'idea che vogliamo investire per pensare un modello anche industriale per territori che tradizionalmente sono zone interne e su cui bisogna pensare in maniera sistemica. Per gli

quell'elemento vitale che resta quando un corpo è debole, che dà la sensazione che da lì possa ripartire la vita. Sopratutto, rappresenta un esempio per coloro che magari sono più fragili e tendono a deprimere le proprie risorse di fronte a una calamità come questa.

periodi, sapendo che non siamo di fronte a una terra che sarà sismicamente stabile: tutta l'Italia è sismicamente instabile ed è sottoposta, anche per i cambiamenti climatici, a possibili devastazioni

valuti positivamente il lavoro della Commissione. Ringrazio nuovamente i Gruppi politici e i componenti della Commissione per il lavoro svolto e ringrazio l'Assemblea per l'attenzione.

Signora Presidente, colleghi, sottosegretaria De Micheli e sottosegretario Pizzetti, ringrazio il relatore per l'ampia illustrazione che consente a me e ad altri di soffermarci solo su alcuni degli aspetti del decreto-legge che andiamo a trattare e dei problemi che andiamo ad affrontare. Il nostro Appennino è una terra di terremoti: terremoti drammatici che si susseguono nel tempo. Ci lasciano respirare per un po', ma poi l'orco torna a gridare, a distruggere e a stroncare splendide esistenze. È arrivato a tradimento il 24 agosto, nel buio della notte, alle ore 3,36, e a tradimento ha colpito quattro Regioni, uccidendo tante, troppe persone. È arrivato di prima mattina, svegliando tante persone, il 30 ottobre, spalmando in un'area vasta tanto dolore e tanta distruzione. Arrivò il 6 aprile, a casa mia, alle ore determinando la fuga, la distruzione e la costatazione della perdita di tante vite umane. Eppure, nonostante il terremoto continui ad arrivare, sembra sempre che non riusciamo a vincere il fatalismo, l'indifferenza o la non convinzione che il terremoto c'è, arriva e, purtroppo, può uccidere.

la risposta dello Stato deve essere ferma, decisa e avvolgente. Così, i due decreti-legge che il Governo ha immediatamente approvato danno risposte forti e importanti. I lavori della Commissione bilancio, che ho potuto seguire grazie alla disponibilità di colleghi che ho potuto sostituire, sono stati proficui e il lavoro di sintesi, non facile, tra i due diversi

Importante è stato il contributo del Governo, di tutti i Capigruppo e di tutti i componenti della Commissione competente. I due decreti-legge, messi a sintesi, danno risposte mature ed avanzate, alcune positivamente sperimentate nel terremoto d'Abruzzo, altre nel terremoto dell'Emilia e altre del tutto innovative. Si fa tesoro di errori, superficialità, impostazioni sbagliate e si superano già, in prima battuta, ostacoli che, ad esempio, nella difficile ricostruzione di L'Aquila solo in questa legislatura abbiamo potuto affrontare e risolvere, grazie anche alla determinazione della sottosegretaria De Micheli e all'ostinazione di tanti di noi e di tanti amministratori. Trovo forte, decisa e coraggiosa la scelta della ricostruzione complessiva. Certo, essa è costosa, ma come si può sottoporre un borgo, nella sua univocità, ad una differenza tra prime e seconde case?

Approfitto di questa occasione per segnalare il problema e per indicare questa, dei decreti-legge del 2016, come la strada maestra per una buona ricostruzione del nostro Appennino. Così facendo, sarà più rapida la predisposizione dei programmi di ricostruzione, la definizione degli aggregati, così come la progettazione organica di questi complessi. Non esito a dire, con carte alla mano, numeri e cifre, con queste regole L'Aquila sarebbe più avanti nella ricostruzione di almeno tre anni. Importanti sono le misure per il rilancio delle attività economiche, la significativa *una tantum* di

sono anche gli ammortizzatori sociali in deroga, la sospensione delle tasse e dei mutui, le positive misure per l'agricoltura, la specifica previsione di un progetto turistico sotto la guida del Ministero competente e l'individuazione delle aree di crisi complessa. Tra l'altro, sono prima firmataria di un disegno di legge che propone nelle aree colpite dal sisma una Zona economica speciale perché queste aree sono anche attraversate dalla presenza di due importanti parchi nazionali, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco nazionale dei Monti Sibillini. Sono aree di grande interesse paesaggistico, sorgenti di straordinaria qualità dei prodotti alimentari, borghi di impianto medievale,

Il cratere o, meglio, i crateri, includono numerosi Comuni in Abruzzo, quattordici, ivi compresa la grande città di Teramo, e poi Campotosto, Montereale e Capitignano, nella Provincia di L'Aquila, e Rocca Santa Maria, Valle Castellana,

L'individuazione, tra l'altro, è stata giustamente fatta di concerto tra Stato e Regione, con un ruolo importante dei vice commissari. Anche questo è da segnalare rispetto alle esperienze passate. È da segnalare anche il fatto che i Comuni e i sindaci hanno poteri diretti e immediati, financo nella scelta delle aree: lontani sono i tempi dei commissari che si sostituivano complessivamente ai poteri locali. Accolgo, quindi, positivamente le tante previsioni. L'Abruzzo però, in questo terremoto, ha subito danni importanti, così come le altre zone,

le procedure di ricostruzione sono ancora *in itinere*. Positivo, quindi, è stato l'accoglimento dell'emendamento che ho proposto che risolve possibili contenziosi e armonizza la legislazione del 2009 con quella del 2016, almeno sulla scelta di quali regole si debbano adottare per la ricostruzione. Ci sono però questioni in sospeso. In uno stesso Comune in Abruzzo, a volte su immobili l'uno a fianco all'altro, si applicano procedure diverse. Ciò che era addirittura reato nel 2009, qui è previsto e, in taluni casi, giustamente incentivato. Allora, dovremo armonizzare. Lo faremo in un altro momento, sono certa che ci sarà disponibilità

Abbiamo dato disponibilità a mettere a disposizione le energie degli uffici speciali, che oggi si occupano delle pratiche di ricostruzione del terremoto 2009, ma la formula individuata inizialmente nel provvedimento è eccessiva (non ci possiamo permettere di allontanare venti persone dalla ricostruzione del cratere 2009); la formula individuata come mediazione la trovo molto ponderata ed equilibrata e mi auguro che domani venga sottoposta all'Assemblea, altrimenti la conseguenza

il lavoro che abbiamo fatto ed è troppo di successo questo strumento, per lasciare in sospeso una piccola cosa per noi però enormemente importante. Ringrazio

che, senza alcuna gratifica materiale, stanno svolgendo un ruolo di guida per popolazioni spaesate e disorientate va sicuramente fatto in quest'Assemblea. saluto le studentesse e gli studenti dell'Università di Bologna, Scuola di giurisprudenza. Benvenute e benvenuti in Senato. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, innanzitutto, diciamolo: in questi giorni più che mai bisogna dire «menomale che il bicameralismo paritario c'è». Avrà le sue storture e criticità,

(cito le comunità di Amatrice, di Accumoli, di Arquata del Tronto, di Norcia e di Cascia), che in più di un'occasione io e alcuni colleghi siamo andati a trovare per capire le loro necessità ed esigenze, il Gruppo della Lega Nord ha dato la massima disponibilità a comprendere, pazientando anche troppo per la presentazione dei decreti-legge (in particolare il secondo), ancora una volta annunciati in pompa magna, con *slide*, da Renzi, ma di fatto resi disponibili con diversi giorni di ritardo. I tempi per la fase emendativa sono risultati molto, troppo compressi. Abbiamo anche rinunciato, nostro malgrado, a segnalare al relatore e al Governo diversi emendamenti che ritenevano meritevoli di attenzione e approvazione. Ci spiace che anche dei pochi emendamenti segnalati tra i diversi presentati, frutto - lo sottolineo - di richieste pervenute dai territori colpiti dal sisma, ci sia stata una sostanziale bocciatura da parte di Governo e maggioranza o al limite l'approvazione di qualche ordine del giorno, che vale poco più di zero. Non ci riteniamo soddisfatti dall'approvazione di pochissimi nostri emendamenti, alla defiscalizzazione delle erogazioni liberali nei confronti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, versati da privati a seguito del sisma, oppure l'emendamento riguardante la possibilità di fare la perizia asseverata in luogo di quella giurata per dimostrare il nesso tra causa ed effetto se uno ha subito danni dal sisma. Nel documento finale, frutto della fusione di due decreti-legge, riteniamo sbagliato blindare il cratere. Per i Comuni che sono stati colpiti e che restano fuori (a quanto pare, tanti) cittadini e imprese non beneficeranno delle provvidenze e dei benefici fiscali e, se hanno subito danni alla propria abitazione o opificio, dovranno dimostrare con perizia il nesso tra causa ed effetto. In merito al cratere, inoltre,

sbagliato non consentire deroghe urbanistiche per l'installazione presso le abitazioni di piccoli manufatti in legno quali luoghi di protezione civile personale per il ricovero immediato in occasione di futuri terremoti e sciami sismici, visto che siamo in aree ad alta ed elevatissima sismicità. Questa è forse la richiesta più invocata da parte di quelle popolazioni, a cui voi state rispondendo no. sbagliato prevedere l'installazione di *container*, acquistati o noleggiati, in pendenza dell'installazione delle strutture abitative di emergenza (SAE), al fine di ovviare agli sfollati di trascorrere l'inverno in tenda senza la dotazione personale di servizi igienici. Bagni e docce saranno comuni. Dunque anziani, disabili e bambini piccoli dovranno, magari di notte, uscire al freddo per i propri bisogni. E intanto apprendiamo che anche la fornitura dei *container* non sarà così veloce e che, anzi, solo pochi manufatti potranno arrivare entro Natale: vuol dire che molti passeranno gran parte dell'inverno in tenda. Con i nostri emendamenti non chiedevamo il *wi-fi*, come pretendono molti sedicenti profughi accolti in albergo, ma almeno *container* con bagni a famiglie con anziani e disabili. È sbagliato non inserire nel testo l'esplicito riferimento alle pertinenze e annessi riferiti all'edifico o all'opificio distrutto o inagibile, che dovrebbero essere rifatti con completo risarcimento dei costi. Nella ricostruzione *post* terremoto dell'Emilia, che non è un esempio di efficienza, relatore Lai (che comunque ringrazio per il lavoro svolto), la mancanza di tali termini nel relativo decreto-legge ha creato una serie di problematiche in quanto non garantiva l'ammissione implicita al contributo e pertanto si è reso necessario emanare apposite ordinanze per definire tali questioni. Bocciare i nostri emendamenti significa non voler tenere conto dell'esperienza del passato e non intervenire per evitare perdite di tempo e i ritardi che hanno caratterizzato la ricostruzione

dove, a fronte di questi "buchi" e di queste criticità, il commissario è già arrivato ad emanare ben 459 ordinanze. Troviamo poi assurdo, anzi gravissimo, che il Governo, in nome di un ambientalismo talebano, in nome dell'efficientamento energetico smisurato e da perseguire a tutti i costi, arrivi a risarcire integralmente i costi di ricostruzione di un edificio con costosissimi interventi interventi innovativi e migliorativi, atti ad esempio a consentire il passaggio da una bassa classe energetica tipo F, o persino G, ad una classe energetica A, e poi non riconosca l'adeguamento sismico degli edifici privati con un livello di sicurezza almeno dell'80 per cento rispetto a quello di un immobile di nuova costruzione.

colpiti in passato e ricostruiti con quei parametri che oggi qui volete riconfermare, sono crollati lo stesso con il ripetersi delle scosse sismiche? Colleghi, quelle zone del centro Italia sono classificate ad elevatissima ed elevata sismicità. Nelle profondità ci sono le faglie, c'è il «mostro», come l'ha definito Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice, che, come la storia più recente dimostra, saranno sempre oggetto, in futuro, di nuovi sismi, contro i quali è necessario Se vogliamo evitare di spendere il doppio di risorse per rifare due volte gli edifici crollati, occorre prendere opportune misure per garantirne la stabilità e il coefficiente dell'80 per cento, che ci avete bocciato, risponde a tale criterio. Qui, colleghi, dobbiamo dare un nuovo ordine alle priorità di intervento da sostenere economicamente con contributi statali: prima, nettamente prima, viene l'adeguamento antisismico che salva immobili, mobili e soprattutto vite umane e poi, se avanza qualcosa, si può pensare anche all'efficientamento energetico *(Applausi prevedere solo la sospensione, e per un tempo limitatissimo (settembre 2016), degli obblighi di versamento delle tasse, dei contributi, dei tributi, delle rate di mutuo, dei premi assicurativi, delle bollette dei servizi a consumo come acqua, energia elettrica, gas, telefono e canone Rai. Bisognava accogliere la nostra proposta di esenzione delle tasse per tre anni, invece niente. Pertanto, famiglie e imprenditori, presto, non solo si ritroveranno costretti a pagare, ma anche a restituire gli arretrati per effetto della sola sospensione. Renzi, come un disco rotto, da settimane, continua a ribadire che per la ricostruzione ci sono i soldi, anche se nei due decreti-legge ne vediamo pochi perché tutto il grosso viene rinviato alle leggi di stabilità, era nell'esenzione delle tasse che doveva dirottare risorse, alleviando le preoccupazioni di cittadini e di imprenditori. Era qui, in questo punto, sull'esenzione delle tasse che doveva fare la voce grossa contro l'Europa. Ci spiace, inoltre, che si sia voluta rinviare la nostra proposta di istituire una zona franca per introdurre agevolazioni fiscali per le microimprese localizzate nei Comuni del cratere. Niente zona franca che, invece, si poteva fare, sottosegretario De Micheli, senza vincolare le risorse. Niente zona franca, ma solo un impegno ad attivarla. Niente esenzioni, con danno a quelle popolazioni senza prospettive, ma solo con un futuro pieno di incertezze. Prima delle conclusioni, desidero, a nome del Gruppo della Lega Nord, ringraziare tutti coloro che si sono prodigati all'indomani del sisma: di quello del 24 agosto, del 26 ottobre e del 30 ottobre. La Protezione civile, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, la Croce rossa, l'ANPAS e i tanti volontari, naturalmente i sindaci in prima linea e porgere un caro saluto alle popolazioni. Il proseguimento della discussione generale e la fase degli emendamenti saranno determinanti per il voto finale del Gruppo Lega Nord e Autonomie.

che, dopo aver pianto le troppe vittime della scossa di agosto, hanno dovuto fronteggiare uno sciame continuo e devastante sino al mattino del 30 ottobre, che ha ridisegnato il profilo del nostro Appennino, ferito lungo quindici chilometri il terreno, aprendo ampie voragini, e riportando in superficie torrenti ormai sotterranei, devastando borghi e comunità, alcune delle quali stavano appena rientrando in un solco di normalità e ripresa economica dopo l'ultimo terremoto del 1997. Borghi interdetti, la cui accessibilità resta La priorità è prestare soccorso e garantire un sistema di gestione dell'emergenza e della ricostruzione, a partire dal ripristino della quotidianità di vita in comune, ripristinare servizi di base a partire dalla scuola, ma anche la ripresa di attività lavorative e di supporto ad una popolazione Popolazione parte della quale ha trovato accoglienza temporanea lungo le coste e, nella mia Umbria, nella zona del lago Trasimeno. Un decreto-legge che opportunamente, come è stato detto, estende l'elenco dei Comuni danneggiati da parte del commissario straordinario, a cui applicare le misure di sostegno al reddito dei

nonché per l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative e anche per le attività produttive, avvalendosi della CONSIP anche attraverso procedure negoziate. Ma un'altra priorità mi preme sottolineare, affinché sì intervenga senza ritardo: il recupero e la salvaguardia di un patrimonio culturale inestimabile, che va dalle tele custodite nelle chiese ormai crollate, ai manoscritti del Leopardi, agli Statuti del Cinquecento, sepolti sotto le macerie delle mura civiche, come a Visso. Dopo il primo intervento dei Vigili del fuoco è necessario subito attivare un piano di recupero, salvaguardia e messa in sicurezza da parte del Ministero, in attesa che diventi operativo l'ufficio speciale della sovrintendenza previsto nel decreto-legge, perché quello che non è riuscito a distruggere il terremoto, potrebbero farlo le condizioni atmosferiche

custode di tradizioni rurali e di una spiritualità religiosa e naturale, di un paesaggio unico; custode di un patrimonio immateriale e culturale che rischia di andare disperso se non riusciremo presto a riportare in quei luoghi i propri abitanti, giovani e anziani. Quella comunità di vita di relazione che parte dal suono della campanella di una scuola o dai rintocchi dei campanili delle torri civiche che scandiscono la quotidianità, ora da ricomporre. Ricostruire in sicurezza, con modelli e regole nuove, come è stato detto, che prospettino ricostruzioni di interi centri storici, tra beni privati e beni del patrimonio pubblico; una ricostruzione a tutela di quella biodiversità, che è al tempo stesso produzione e trasformazione di qualità di prodotti tipici di marchio IGP e DOC DOC (dallo zafferano, alle lenticchie, ai tartufi, ai formaggi), di luoghi un tempo affollati di turisti che in quei posti andavano per gustare il silenzio, i sapori e gli odori, attratti dalla bellezza dell'autenticità dei luoghi e delle loro tradizioni irriproducibili e uniche. Sono borghi che spesso sono stati di pubblicità ideali di prodotti quali quelli dell'azienda Perugina, che di recente ha dichiarato il suo impegno per la ricostruzione e la rinascita di Castelluccio; ma vanno ricordati anche altri privati, come Brunello Cucinelli, che ha dichiarato ha dichiarato il suo impegno in favore del monastero dei benedettini di Norcia. Penso ad un patto per il territorio tra pubblico e privato, per questo sosteniamo la posizione assunta dal nostro Governo affinché la Commissione europea e i Paesi membri riconoscano e concedano la flessibilità nei conti nazionali per le spese necessarie per la gestione dell'emergenza, ma anche per la ricostruzione, per la messa in sicurezza degli edifici, in una prospettiva di un piano Casa Italia che rappresenti in concreto un'opportunità di valorizzazione un Paese straordinario, percorso però da tante fragilità, ma che ancora oggi, come ha detto il relatore, manca di un sistema predefinito di poteri e di *governance* utile per la gestione delle emergenze, un sistema predefinito, snello efficace e al tempo stesso chiaro e trasparente. Questo potrebbe essere l'impegno che oggi si assume il Parlamento, per dare chiusura e completamento al sistema creato con la legge del 1992; in maniera automatica, con compiti, poteri e strutture funzionali; un sistema non permanente, straordinario, ma in grado di attivarsi senza dover aspettare un decreto-legge da convertire. un sistema di poteri commissariali che valorizzi anche Protezione civile, Vigili del fuoco, forze di polizia e tutto il volontariato che è intervenuto a prestare i primi soccorsi e che da lì non se ne è mai andato ed è restato accanto ai sindaci. Da Amatrice a Norcia, con la sua basilica, rappresentino per tutti noi il campo di prova della capacità di un popolo che non si arrende di rilanciare quei luoghi, simbolo e storia di forza spirituale e materiale, terre da far rifiorire.

tanta angoscia da parte dei nostri concittadini. Io ho ancora vivo negli occhi il ricordo delle prime immagini viste nei giorni successivi alla scossa che colpì Amatrice, quando, insieme al senatore Arrigoni, ci recammo nelle zone terremotate, e ancora più vivo ho negli occhi l'immagine delle stesse zone, visitate di nuovo solamente la scorsa settimana, con i paesi irriconoscibili,

In Commissione sono stati fatti approfondimenti importanti, il relatore ne è stato sicuramente all'altezza e da parte di tutti i Gruppi c'è stata una volontà molto importante, in termini proprio di condivisione delle scelte. Non Non mi è piaciuto vedere un atteggiamento del Governo essenzialmente improntato ad asciugare le proposte dei Gruppi di opposizione per farle apparire assorbite, per dimostrare che l'azione fatta dal Governo con il provvedimento è di per sé sufficiente a dare le risposte.

piccole o singole, ma valevano per categorie generali come dare una risposta abitativa, come dare una risposta all'emergenza, come dare una risposta all'angoscia di chi viene colpito dal terremoto.

Viene descritta dalle televisioni un'azione di Governo con grande dispendio di risorse e di energie, ma basta andare nella palestra di Cascia e vedere - come abbiamo visto noi nei giorni scorsi - gli anziani radunati, annientati nella loro capacità anche di guardare ad una prospettiva. Basta vedere le code delle persone per avere un piatto di pasta, in una giornata peraltro non brutta, senza copertura. Questi sono gli aspetti su cui abbiamo chiesto e avremmo voluto avere delle risposte più aderenti alla realtà.

a esempi di sciacallaggio sui terremoti passati, con chi si è approfittato delle disgrazie per arricchirsi, però non per questo bisogna mettere in secondo piano

di un tessuto abitativo che è fatto da persone e non solo da case e strutture. Signora Presidente, se lei va a Norcia, si accorgerà che ci sono attività

persone che sono lì, senza avere una struttura nella quale poter continuare a essere residenti. Quando i pullman hanno prelevato le persone da Norcia e dagli altri Comuni della Valnerina e le hanno ho parlato con persone che realmente si sono sentite deportate, perché sono state prese, caricate sui pullman e scaricate le sera stessa in alberghi e residence senza avere a disposizione nulla:

E rispetto a questa realtà, purtroppo, vi è stato un desiderio di non approfondire. Abbiamo proposto emendamenti piccoli, semplici, anche a valere sui Comuni che considerare che quelle sono zone in cui il terremoto si ripresenta costantemente e dove purtroppo gli intralci posti in mezzo, una volta dai beni ambientali, una volta una volta dal parco, una volta dalla burocrazia, hanno impedito anche la costruzione di piccoli presidi di tutela e salvaguardia, che invece avrebbero consentito e consentirebbero alle persone, nel momento in cui si presenta una scossa di terremoto,

e il Governo dice che, alla fine, è talmente complessa la materia che la vedremo la prossima volta, perché bisogna metterla a fuoco. Ma cosa volete mettere a fuoco? Andate a parlare con la gente, con i sindaci. Confrontatevi con il territorio, e non solo con i funzionari della Protezione civile.

si valuta la maturità dell'azione politica. Avete chiesto alle opposizioni di non fare attività di ostruzione e non è stata fatta, perché non poteva essercene su un tema così importante. Vi abbiamo proposto correzioni che in qualche caso vi evitano e vi hanno evitato, come eviteranno ai cittadini, di fare una perizia giurata anziché una perizia asseverata, evitando di mandare i propri tecnici a fare burocrazia in Comune e in tribunale per avere la certezza che la casa, invece, è crollata, quando è lì da vedere.

di sapere che c'è anche la possibilità di fare attività e di creare economia; altrimenti, cosa si ricostruiscono a fare le case, se poi non c'è nessuno che potrà abitarci perché non c'è un'economia che li sostiene? PRESIDENTE. C'è l'amarezza, signora Presidente, di non aver visto considerare tutto questo, con un atteggiamento che credo abbia fatto leva su un ricatto morale: non potete fare opposizione, non potete insistere troppo sugli emendamenti perché non potete dire di no a un decreto-legge che riguarda il terremoto.

Consiglio dei ministri: avete chiesto di trasformare gli emendamenti in ordini del giorno e di ridurre gli ordini del giorno in raccomandazioni. Siate seri:

*(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, le parole che dal 24 agosto ad oggi ho sentito pronunciare con maggiore frequenza da coloro che hanno vissuto sulla propria pelle la terribile esperienza del sisma sono: «Non ci lasciate soli!». In effetti siamo ormai consapevoli che, anche in occasione di eventi che scuotono profondamente le nostre sensibilità, le luci del circo mediatico si accendono improvvisamente e ancor più velocemente sono destinate a spegnersi. Ma, al di là dell'attenzione effimera dei mezzi di informazione, abbiamo il dovere, come rappresentanti delle istituzioni, di ascoltare questo appello, che trova piena legittimità nell'aspettativa di ricevere un aiuto a risollevarsi dopo il colpo durissimo inferto dal terremoto. La situazione che ho avuto modo di constatare testimonia con forza ancora oggi che siamo di fronte a qualcosa di eccezionale. La vicinanza che le persone colpite chiedono è legittimata anche dall'insostenibile condizione psicologica che si trovano ad affrontare quotidianamente, nel tentativo di ritornare alla normalità e nel convivere con i fenomeni sismici che tuttora persistono: uno stillicidio sismico che ad oggi ha sviluppato 25.000 scosse, di cui oltre 300 superiori al 3° grado. del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il cuore dell'Italia, interessando un area di oltre 600 chilometri quadrati provocando ingenti danni ai 131 Comuni di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio che costituiscono il cosiddetto cratere; un evento distruttivo che ha coinvolto 300.000 persone e provocato danni a oltre 200.000 edifici. Alla Provincia di Macerata, che si è vista risparmiare le vittime (se non in un singolo caso), sono stati però riservati i danni più rilevanti: 46 Comuni, sui 57 complessivi che compongono la Provincia, rientrano nel cratere; molti i municipi inagibili, 37 le scuole inagibili e quasi 25.000 sono le persone, delle 30.000 complessivamente assistite, nell'ambito del territorio della Provincia di Macerata. Non è migliore il quadro delle attività produttive, dove 917 strutture sono inagibili (rappresentano circa l'80 per cento del totale); così come nella zootecnia, dove 110 stalle sono inagibili (quasi la metà del totale Il provvedimento all'esame in questo senso appare all'altezza dell'impegnativa sfida da affrontare, un primo passo concreto per superare l'emergenza e avviare la ricostruzione. Per l'enorme e straordinario lavoro che è stato messo in atto, per la tempestività e spero anche per la condivisione con cui quest'Aula approverà il provvedimento, voglio ringraziare tutti coloro che si sono dedicati alla stesura, alla correzione e all'integrazione di tale documento e, per tutti, il collega relatore Silvio Lai. Delle tante misure che il decreto-legge introduce mi limito a citare alcune tra le più rappresentative: la risarcibilità integrale dei danni delle seconde case ricomprese nel cratere del sisma e anche all'esterno, nel caso di centri storici e borghi caratteristici, riconoscendo con ciò che in questi territori le seconde case sono abitazioni di famiglia e prezioso fattore di sopravvivenza dell'economia locale; le misure rivolte sia a far ripartire le imprese esistenti, sia a crearne di nuove, e quelle a tutela dei lavoratori; la semplificazione amministrativa rivolta a facilitare i lavori per riparare in tempi brevi le case lievemente danneggiate. È evidente a tutti come, in una situazione così estesa e perdurante, non possa esserci in questo provvedimento tutto ciò che sarebbe auspicabile. Esso contiene, però, tutto ciò che appare necessario in questa fase. E vorrei sottolinearne il valore anche in relazione al fatto che esso non si occupa solo di ricostruzione edilizia, ma anche di economia, di turismo e cultura. In realtà, nei 131 Comuni colpiti il problema non sarà ripristinare la situazione precedente al sisma, ma invertire una tendenza allo spopolamento e all'abbandono che, negli scorsi anni e decenni, ha colpito molti dei piccolissimi Comuni coinvolti. lo si farà promuovendo politiche di sviluppo incentrate sui punti di forza di questi territori che sono la natura e il paesaggio, le produzioni agricole e agroalimentari specializzate, il turismo, il patrimonio culturale e le produzioni manifatturiere artigianali. Anche per queste ragioni è importante - e il Governo ne ha assunto l'impegno - rispettare l'identità dei luoghi e degli edifici, salvaguardando così l'identità e l'integrità dei centri abitati e delle comunità. È ovvio che un tale compito chiami in causa una strategia che va oltre i confini del provvedimento in esame e che deve pienamente coinvolgere altri strumenti normativi, - la legge sui piccoli Comuni, in discussione in quest'Aula nei prossimi giorni, e la strategia delle aree interne: tutti strumenti che devono concorrere in modo coerente al perseguimento degli obiettivi prefissati e al rilancio di questa parte d'Italia. Negli oltre 600 chilometri quadrati colpiti dal sisma ricadono due parchi nazionali - quello dei Monti Sibillini e quello del Gran Sasso e Monti Laga - attraverso i quali la tutela dei valori ambientali può essere messa al servizio della rinascita di queste aree. Anche la nuova legge sulle aree protette, recentemente licenziata dal Senato, offre strumenti e opportunità per un ruolo attivo dei parchi in tale direzione e proprio il sindaco di uno dei Comuni più colpiti, il sindaco Rinaldi di Ussita, nei giorni scorsi ha definito questa norma importante e significativa per il riscatto del territorio. Gli eventi sismici hanno colpito e sferrato un duro colpo a due delle più antiche università del nostro paese - e l'università di Macerata e Camerino rappresentano una comunità di 20.000 studenti. Se l'ateneo di Macerata ha subito minori ma non marginali danni, per Camerino la situazione è davvero drammatica. 30.000 i metri quadri di superfici inagibili, 1.000 gli studenti che necessitano di una abitazione e altri 500 residenti tra Marche e Umbria che, dopo un periodo di pendolarismo, avranno l'esigenza di una stabilità abitativa. L'ateneo di Camerino, in particolare, anche in virtù della sua collocazione geografica, è un solidissimo punto di riferimento di tutto l'entroterra alto collinare e montano delle Marche. Già precedentemente al sisma esso rappresentava un motore di sviluppo per le piccole medie imprese e per gli enti del territorio quanto a promozione e valorizzazione delle eccellenze manifatturiere, enogastronomiche, turistiche e tecnologiche. Proprio da questa situazione emergenziale potrebbe nascere dall'università di Camerino un polo scientifico-tecnologico di riferimento a supporto delle imprese e della pubblica amministrazione. l'ateneo ha già da tempo richiesto la cessione dell'ex presidio militare delle «Casermette» al Ministero della difesa in quanto bene del demanio. Anche l'università di Macerata, con la sua caratterizzazione umanistica, diventare, nella fase di ricostruzione, punto di riferimento offrendo personale qualificato nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio artistico diffuso sul territorio.

Sarà indispensabile una implementazione delle risorse, perché dobbiamo pensare che le aziende non torneranno a produrre reddito nel breve periodo e i flussi turistici subiranno una forte contrazione per un periodo molto lungo. quindi, un lavoro incessante per garantire l'efficienza e l'efficacia della ricostruzione. Il passaggio dall'emergenza alla ricostruzione evidenzia complessità e difficoltà che dobbiamo affrontare, a partire da una tempestiva attivazione e corretta distribuzione sul territorio degli uffici speciali per la ricostruzione. Non mancano segnali incoraggianti di una forte volontà di rinascita coerenti con la tempra di un popolo abituato a misurarsi con grandi fatiche e difficoltà quotidiane.

A Gualdo, lo scorso fine settimana, è stata inaugurata una nuova scuola costruita a tempo di *record*, in tre settimane. A Visso ha ripreso l'attività, proprio in questi giorni, la Svila, una importante azienda *leader* nella produzione di La vera spinta propulsiva di questi segnali di risveglio sono i sindaci, la più alta espressione della tenace volontà di difendere e garantire un futuro alle comunità rappresentate: il loro infaticabile e generoso operato serve a riscattare non solo le sorti della propria gente, ma anche quelle di una politica troppo spesso oggetto di scherno. Occorre comunque dire che tutti i livelli istituzionali coinvolti nella fase emergenziale hanno garantito, insieme al volontariato, alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco e alle Forze dell'ordine, un impegno all' altezza della situazione. sottolineando in particolare l'impegno e il ruolo del commissario Errani. In conclusione, riprendendo l'appello «Non lasciateci soli», non possiamo trascurare che i valori ambientali, culturali, artistici e i saperi locali, di cui quei territori sono custodi,

Saluto la delegazione dell'associazione dei giovani e delle giovani amiche dei musei d'Italia, cui do il benvenuto in Senato.

la situazione che stanno vivendo gli abitanti delle aree colpite dal sisma del 24 agosto e del 26 ottobre richiede grande attenzione per le dimensioni che si sono registrate, ma soprattutto richiede di intervenire con urgenza. La macchina che si è messa il moto per la prima emergenza ha potuto contare sull'importante supporto della Protezione civile, diventata negli ultimi anni, a seguito dell'abolizione della leva militare, una vera e propria risorsa umana. Prezioso è il lavoro dei Vigili del fuoco, che vedono impiegate circa 1.500 unità, e delle altre Forze dell'ordine. In questa occasione l'Italia ha dimostrato di essere unita nel lutto, ma anche nel desiderio di far ripartire quei luoghi. Superata la fase della prima emergenza, è necessario ora guardare a interventi strutturali che consentano *in loco* una soluzione abitativa per gli sfollati, che, dimostrando grande attaccamento alla propria terra, chiedono giustamente di essere messi nelle condizioni di restare nei loro paesi. C'è necessità quindi di una *governance* innovativa rispetto a quella attuata in occasione di precedenti eventi sismici, che già dalla prima fase si proietti nel futuro con la finalità di ricostruire mantenendo l'identità territoriale e la cultura del luogo. Con questo intervento mi limito ad affrontare due argomenti di competenza della 7ª Commissione, di cui faccio parte: in questa ottica è importante che il provvedimento in esame introduca alcune norme derogatorie per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017, tenuto conto dell'elevato numero di istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati (224) e degli edifici scolastici (circa 450); la popolazione scolastica coinvolta è di alcune decine di migliaia di alunni. È da accogliere con soddisfazione che la maggior parte degli alunni e studenti abbia potuto riprendere le lezioni: in alcuni casi solo pochi giorni dopo il secondo sisma; in altri con tempistiche dilazionate e più lunghe (proprio ieri per alcuni studenti del liceo). Il decreto-legge prevede la possibilità di derogare ai parametri minimi e massimi per la formazione delle sezioni e delle classi; l'istituzione di ulteriori posti di organico, di natura temporanea, sino al 30 giugno 2017; lo spostamento di docenti, a seguito di contratto integrativo regionale, tra le sedi scolastiche. La flessibilità della norma prevista dal Governo sul numero minimo di alunni per classe e sul reclutamento dei docenti va nella giusta direzione di favorire la permanenza della popolazione - in questo caso quella scolastica - nei propri paesi. Far capire fin da subito, in particolare ai giovani e agli studenti, che la soluzione a cui guardano il Governo e le comunità locali è proprio quella da loro auspicata che garantisca la permanenza ha sicuramente anche un effetto psicologico nel percorso per superare il trauma subito. Ma con questo intervento voglio sottolineare anche un altro aspetto: il sisma verificatosi ha richiamato l'attenzione sul grandissimo patrimonio monumentale, artistico e ambientale presente in quei luoghi; un patrimonio che richiama origini antiche, una storia lunga secoli, ma anche il forte radicamento dei residenti in quei borghi, molti di dimensioni limitate, in cui il persistere di tradizioni e occupazioni antiche si coniuga con la modernità. Nei territori colpiti ricadono anche due parchi nazionali e diverse aree soggette a misure di salvaguardia, ai sensi della vigente legislazione in materia paesaggistica: un patrimonio che ha subito lesioni gravi, che rischiano di portarlo al dissolvimento. Appare quindi necessario affrontare con determinazione il tema della messa in sicurezza dal punto di vista sismico e del recupero della tutela del paesaggio e dei beni culturali esistenti.

questa la sede per disquisire sulle modalità di intervento: il decreto-legge affida a chi ha responsabilità amministrative e competenze tecniche tale compito. Fondamentale è comunque aver previsto procedure più snelle e veloci per assicurare che gli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione perseguano sempre il massimo grado di compatibilità con le esigenze di conservazione e salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali esistenti. In questi luoghi, peraltro, l'ambiente e il paesaggio costituiscono una risorsa da valorizzare in sé ai fini del rilancio dell'economia locale, che, storicamente, ha nel turismo una prerogativa di assoluta importanza. Al fine di disporre di maggiori risorse e per accelerare il processo di ricostruzione, è importante la previsione di fare ricorso al credito di imposta previsto dal decreto-legge n. *art bonus*, anche per le erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso, presenti nei Comuni e di proprietà non pubblica.

decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Innanzitutto desidero rivolgere un ricordo a tutte le popolazioni colpite dal terremoto, che hanno perso i propri cari, le proprie case e i propri averi. Non possiamo lasciare che i rancori tra le compagini politiche possano mettere in discussione la coesione e la solidarietà. Dobbiamo rimanere uniti ai nostri connazionali, alle forze armate e ai civili impegnati sul campo. Ormai sono passati tre mesi da quel terribile 24 agosto e meno di un mese dagli ultimi tragici eventi. L'atteggiamento tenuto dal Gruppo di Forza Italia è stato sempre volto alla collaborazione con il Governo e con tutte le autorità per l'opera di emergenza e di ricostruzione delle aree colpite. Il Governo Renzi, invece, è stato ostile al dialogo e mi accingo a spiegarvi perché. Il giorno 28 agosto dichiarato che avrebbe coinvolto il Parlamento e le opposizioni in tutte le discussioni in merito al sisma avvenuto nel Centro Italia. Disse che avrebbe preso in considerazione tutte le parti politiche, ma purtroppo questo non è accaduto. È venuto meno il confronto, anche per la nomina politica del commissario straordinario Vasco Errani, mentre avrebbe dovuto essere una figura tecnica *super partes*. Non è mai opportuno fare dei parallelismi quando si mettono a confronto eventi catastrofici di questo tipo, ma mi trovo costretta a farli e a sottolineare l'atteggiamento inopportuno del Governo Renzi di fronte al sisma che si è abbattuto sull'Italia centrale. Il primo decreto-legge è stato presentato il 17 ottobre 2016, quasi due mesi dopo i tragici eventi sismici. Avvenne il contrario durante il Governo Berlusconi, con il terremoto che colpì l'Aquila e l'Abruzzo nel 2009. Il comportamento tenuto dal centrosinistra fu polemico e avverso nei confronti di ogni singola azione che il Governo Berlusconi decise di attuare; un atteggiamento pessimo e disdicevole in quel frangente. Il Governo Berlusconi deliberò il primo decreto-legge in favore dei Comuni colpiti dal sisma il 28 aprile 2009 e il sisma si verificò il 6 aprile, dopo soli ventidue giorni. I risultati dell'intervento immediato sul territorio abruzzese sono ancora oggi sotto gli occhi di tutto il mondo. Nel settembre del 2009, circa 35.000 «sfollati» ebbero accesso ai moduli abitativi provvisori (MAP) e, in seguito, ci fu l'attuazione del progetto CASE, le case antisismiche definitive. Il Governo Renzi parla di *container* da consegnare alle popolazioni colpite dal sisma a tre mesi dal verificarsi delle prime forti scosse. L'inverno è alle porte; le avverse condizioni climatiche sono un problema per le persone che hanno deciso di non abbandonare il proprio territorio e il ritardo e l'inadeguatezza della «macchina di pronto intervento» sono destinati a far pagare loro le conseguenze, qualora non ci sia una immediata inversione di tendenza. In questa circostanza le opposizioni attuali non hanno adottato lo stesso atteggiamento polemico e poco costruttivo fatto proprio dalla minoranza parlamentare di allora. Nonostante tutto, siamo qui come Gruppo Forza Italia a collaborare in pieno in modo efficace per la realizzazione di una legge che tuteli e intervenga con efficacia in tutti i territori colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre di quest'anno. Il maxiemendamento del Governo al decreto-legge assorbe largamente anche i contenuti del decreto-legge n. 205, recante i nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni, ed estende le disposizioni anche ai territori interessati dagli ultimi eventi sismici. Il secondo elenco dei Comuni si unisce al primo, ampliando l'elenco di quelli che entrano nel cratere sismico. Vengono introdotte norme speciali per le strutture e i moduli abitativi provvisori, che verranno rimossi alla cessazione dello stato d'emergenza. Va evidenziato, inoltre, che i territori colpiti sono ricchi di un patrimonio artistico-culturale unico al mondo, della cui ricostruzione devono farsi carico anche l'Europa e il mondo intero. Su questo serve una forte azione diplomatica nelle sedi internazionali. L'Italia però dovrà farsi carico della ricostruzione degli immobili e della continuazione delle attività economiche. Per fare queste cose servono risorse importanti che ancora non sono previste nei due decreti-legge, ora assorbiti nel decreto-legge Non vanno dimenticati i bambini e i giovani, i quali hanno diritto al ritorno alla normalità e alla spensieratezza dell'età che portano. Soprattutto a loro dobbiamo dare una speranza e la certezza che possano tornare alla vita di prima. In conclusione, auspico che, dopo gli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia quest'anno, si applichino interventi strutturali preventivi per la riduzione del rischio sismico. Anche per questo servono opportune risorse economiche e spazi finanziari nei bilanci degli enti territoriali, che al momento risultano essere ancora insufficienti. Tutta la fascia appenninica è fortemente soggetta a fenomeni sismici di medio-alta intensità. Questo ci deve mettere davanti alla realtà che tutta la zona - e non solo quella - deve essere messa nella condizione di prevenire e affrontare in sicurezza eventuali nuove tragedie. Mi auguro che ogni famiglia colpita dal sisma possa riavere ciò che ha perso, anche se non sarà mai abbastanza per colmare la tragedia e la paura vissuta. Ma la speranza deve essere suffragata dai fatti, dalla velocità delle decisioni, dalla certezza degli stanziamenti economici che questo decreto-legge, ancora troppo macchinoso e burocratizzato, non sembra ancora dare alle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia.

Non si può parlare di approssimazione in siffatto modo. Non si può dire che in una situazione come questa la Protezione civile non sia stata all'altezza. Solo una vergogna e un'offesa nei confronti di tutti coloro - dal Governo, alle forze di polizia, alle Forze dell'ordine, ai volontari e ai cittadini - che nelle ultime settimane hanno dato una mano, senza fare le sfilate

Non si fa una cosa del genere su quanto accaduto e su una calamità come quella che ha colpito le nostre città. Bisogna essere seri, anche in questo momento. E la serietà vuole che si lavori tutti insieme e si provi a migliorare quello che c'è di migliorabile; che si seguano le cose anche dopo la conversione di questo decreto-legge, ma che si rispetti

Signora Presidente, colleghi, siamo tutti riuniti in quest'Aula per la conversione in legge di due decreti‑legge integrati recanti interventi urgenti e necessari per far fronte alle urgenze dovute al verificarsi dei gravissimi eventi sismici che hanno colpito l'Appennino centrale, coinvolgendo i territori e le popolazioni di ben quattro Regioni: la mia terra d'origine, le Marche, assieme all'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo, e gente laboriosa, dignitosa, umile senza essere modesta, perché ricca di storia, di tradizioni, di sapere e di un passato che abbiamo il dovere di preservare per il futuro, agendo al meglio in questo difficile presente. Sono gli occhi di chi ha avuto modo di visitare i luoghi a narrarci quanto è accaduto. Le immagini sostituiscono le parole e, tra queste, gli sguardi impauriti e smarriti alla ricerca di una casa di una casa che non c'è più, di una normalità svanita, degli oggetti di uso quotidiano, delle cose più care, seppellite tra le macerie; talora di un futuro che non si riesce a immaginare e di un presente al quale non ci si arrende, perché la terra che trema è la stessa che non si vuole e spesso non si può abbandonare, come non si abbandona un familiare fragile o malato, come non si sarebbe voluto perdere degli affetti. Molto è stato fatto per intervenire con urgenza - forse non subito e non ancora tutto per consentire alla cittadinanza di recuperare una minima condizione di normalità, necessaria per nutrire speranza nel futuro senza abbandonare la propria dimensione di affettività e smarrire la propria identità. Noi siamo i nostri luoghi, le nostre abitudini, le nostre tradizioni, le nostre amicizie, la nostra famiglia, il nostro lavoro, e tutto questo dobbiamo difendere e tutelare. Apparteniamo alla città, al paese, al borgo, persino alla via in cui abitiamo, e ne siamo un riflesso vivente, nel bene e nel male, consapevolmente o inconsapevolmente. Ecco perché siffatti eventi non lesionano solo le cose materiali, non ci danneggiano solo economicamente, ma feriscono l'anima con cicatrici indelebili. Quei luoghi conservano passioni, speranze, impegni, impronte di vissuto. Ed è per questo motivo che dobbiamo impegnarci con velocità, efficienza, umanità, serietà e responsabilità. Commovente ed esemplare, a questo proposito, è stata la risposta che è giunta dall'intero Paese, mobilitato in favore delle popolazioni messe in ginocchio dal "mostro", dando un esempio di solidarietà e di comprensione profonda di quanto accaduto. Penso a una grande azienda a Tolentino che ha retto al sisma, e anche questa volta è stata esempio di umanità e pragmatismo, ospitando i terzisti nei suoi spazi, allestendo e ampliando l'asilo anche per i lavoratori di ditte esterne. tutte le istituzioni coinvolte proseguano nell'attuale opera di coordinamento e collaborazione per superare al più presto la fase dell'emergenza e iniziare quella della ricostruzione morale e materiale, di persone e territori. Il sisma si è esteso su un'area molto vasta sconvolgendo oltre 130 Comuni, determinando circa 40.000 sfollati e tantissime - ancora da quantificare e valutare - case danneggiate. Per questo motivo, per lavorare congiuntamente, senza steccati e confini ideologici, mi sono fatto promotrice di un intergruppo bicamerale per il sostegno alle popolazioni nella fase immediata e per la successiva messa in sicurezza dell'intero sistema Paese. Ciò mi sembra una modalità efficace per intervenire trasversalmente in modo concreto e diretto. Invito quindi tutti voi, interessati al governo dell'emergenza e soprattutto alla ricostruzione delle infrastrutture fisiche e morali del nostro bel Paese, iscrivervi a questo intergruppo, e colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente i numerosi che lo hanno già fatto. L'Italia è un Paese geologicamente giovanissimo, anche se culturalmente molto antico, tanto da vantare la presenza della più alta concentrazione mondiale di beni culturali. E di questo patrimonio dobbiamo, non solo essere fieri, ma possidenti passeggeri, leggeri, capaci di agire responsabilmente per tramandarlo alle future generazioni. Un'Italia che il sisma ha spaccato, determinando letteralmente lo spostamento di intere aree geografiche, deve rimanere unita e programmare un futuro diverso, perché fenomeni endemici del nostro territorio, come i nostri terremoti, non possono più portare con sé lutti e rovine. Per questo motivo, il sisma deve essere l'occasione da non perdere per una ristrutturazione dei centri abitati: tutti, dai piccoli borghi alle città metropolitane, realizzando un'anagrafe pubblica degli edifici per conoscere quelli che hanno necessità di interventi preventivi (oggi a rischio più di ieri, perché gli insulti cumulativi delle tantissime scosse non li hanno lasciati illesi), per riqualificare l'ambiente ovunque sia necessario per compiere un'opera di salvaguardia e scongiurare in futuro, per quanto possibile, danni evitabili. I primi interventi prestati alle popolazioni sono stati veloci, compatibilmente con le difficoltà ambientali che hanno dovuto incontrare gli operatori delle forze impiegate per prestare soccorso, a causa della natura montuosa e impervia dei luoghi colpiti dal sisma. L'aver dichiarato immediatamente lo stato di emergenza ha consentito di ottenere risultati celeri. A causa del progressivo allargamento dell'area territoriale, causato causato dal susseguirsi dei numerosi terremoti, vi sono state incertezze e preoccupazioni nell'individuazione dei Comuni compresi nel cratere sismico, cioè quelli che hanno diritto alla ricostruzione A questo riguardo, ho seguito in modo particolare l'evoluzione della situazione dei Comuni delle Marche, sono felice per l'inserimento nel cratere

di snellire le procedure burocratiche a quella di allestire le squadre in modo che la valutazione sia la più obiettiva, la più veloce e la più esauriente possibile e si possa poi ricostruire. Rivolgo un ringraziamento particolare all'ingegner Curcio, della Protezione civile, che, sollecitato a velocizzare le valutazioni della squadre che avevano difficoltà, ha risposto tempestivamente, in giornata, così da avviare poi le schede Fast, che hanno ampliato la platea dei valutatori. Questo è sicuramente importante e ancora di più, forse, si può fare. Questo terremoto ci darà molti più problemi, perché ancora non è stato compreso.

ci sono persone che non hanno più una casa. C'è un problema di abbandono scolastico e di alcuni ragazzi che sono stati dislocati molto lontano. Io ho parlato con il sindaco di Camerino, che è preoccupatissimo, perché, se i figli vanno fuori, i genitori seguono i figli. Egli ha dunque paura dello spopolamento di quelle aree, una paura legittima. Si sono creati dei comitati di cittadini, di mamme, preoccupate per la sicurezza scolastica, in questo risvegliando anche la partecipazione concreta e propositiva di tutti in modo molto positivo.

citando le parole di uno scienziato che ha dedicato la sua vita allo studio dei terremoti, Giuseppe Mercalli, nella speranza che sia giunto il momento di ascoltare queste parole e di tradurle in opere: «La sismologia non sa dire non sa dire quando, ma sa dire dove avverranno terremoti rovinosi e sa pure graduare la sismicità delle diverse province italiane, quindi saprebbe indicare al Governo dove sarebbero necessari regolamenti edilizi più e dove meno rigorosi, senza aspettare che prima il terremoto distrugga quei paesi che si vogliono salvare». Signora Presidente, come è stato riconosciuto dal relatore stesso, le opposizioni hanno avuto un atteggiamento profondamente costruttivo nell'affrontare un decreto-legge così importante per tutte le popolazioni colpite mi dispiace aver sentito pochi minuti fa interventi con toni decisamente accesi e inappropriati in relazione a questa tragica vicenda. Purtroppo non sono stati accolti molti emendamenti migliorativi proposti dalle opposizioni. Lo stesso atteggiamento costruttivo è stato dimostrato in 12a Commissione, alla quale ho l'onore di appartenere, nell'approvare all'unanimità il parere espresso dalla senatrice Dirindin; un parere parere che metteva una condizione fondamentale per la sua approvazione, ovvero quella di inserire nell'ambito dell'articolo 14 interventi strutturali sugli ospedali e sulle strutture sanitarie e sociosanitarie con lo stanziamento di fondi specifici per il quinquennio 2017-2021. È indubbio, infatti, che le strutture ospedaliere, sanitarie e sociosanitarie collocate nelle zone a rischio sismico 1 e 2 posseggano tutte le caratteristiche di edifici di interesse strategico, la cui funzionalità durante eventi sismici assume un rilievo fondamentale. Gli ospedali sono proprio luoghi cui si rivolgono le persone in difficoltà per trovare non solo aiuto e cure, ma anche riparo dai rischi esterni. Mi appello quindi al Governo, a nome del Gruppo di Forza Italia e di tutti componenti della 12ª Commissione, affinché si rivedano nell'articolo 14 gli interventi strutturali sugli ospedali e

la terra ha ripreso a tremare e continua tutt'ora uno sciame sismico, quello del Centro Italia, che inevitabilmente ci porta alla mente la scossa di terremoto del 6 aprile 2009 che a L'Aquila fece 309 vittime, 1.500 feriti, danni per oltre 10 miliardi di euro e più di 60.000 sfollati; ovviamente ci riporta alla mente anche le scosse dell'Emilia-Romagna del 20 e del 29 maggio 2012, con 27 vittime e poco meno di 13 miliardi di danni. Per quest'ultima emergenza per le zone colpite dal sisma finalmente il Governo ha fatto tesoro delle bruttissime esperienze precedenti, non ricominciando dal nulla a scrivere i decreti-legge, ma riuscendo a scrivere un atto abbastanza completo, ma ovviamente ci sono delle criticità. La prima interviene senz'altro sul piano delle coperture, di cui però in quest'Aula si è già parlato e di cui parleranno anche i miei colleghi; l'altra criticità concerne la ricostruzione,

Per non parlare, poi, dei tempi lunghissimi della burocrazia per i troppi ricorsi al TAR. Anche per quanto riguarda la ricostruzione privata, vediamo comunque che solo l'80 per cento dei nuovi quartieri

Come non ricordare il palazzo del Comune e della prefettura e le foto delle macerie che hanno fatto il giro del mondo. Ma è nelle sessanta frazioni di L'Aquila, quelle in cui abitano i cittadini semplici, che vivono di agricoltura e allevamento del bestiame, come le zone colpite da quest'ultimo sisma, che si contano i ritardi peggiori e anche il disagio tra le popolazioni non diminuisce. Mentre la ricostruzione in Emilia-Romagna per il terremoto del 2012 procede più spedita per quel che riguarda le case private, per quanto riguarda il patrimonio pubblico e monumentale viaggia su un binario sempre più lento. Progetti di complessità maggiore sicuramente, ma edifici di pregio architettonico e piccoli Comuni con minore disponibilità di tecnici hanno fatto sì che tutto marciasse a questa velocità più bassa. Il punto debole, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione dei beni architettonici, sembra la dotazione di personale della sovrintendenza regionale, che è troppo scarso per smaltire l'enorme mole di lavoro maturato in questi mesi con il vaglio dei progetti e le verifiche sulla loro attuazione.

Visto tutto questo, in questi decreti-legge è comunque stato previsto un aumento di personale per i Comuni, ovviamente per ovviare ai ritardi, e speriamo che questo personale basti per fare una ricostruzione più veloce. Ma il faro che deve rimanere acceso non è tanto sulle questioni burocratiche, che sono quasi state risolte all'interno del decreto-legge con l'aumento, appunto, del personale: deve rimanere acceso soprattutto per quanto riguarda le associazioni malavitose. Non possiamo dimenticare che a L'Aquila

ma pochi condannati (solo una manciata di imputati) e, poi, alla fine, la prescrizione, problema tuttora non risolto da questo Governo. In tal senso, non è meno critica la situazione nelle aree della Bassa emiliana colpite dal terremoto del 2012. Il tanto decantato modello Emilia, che, secondo la narrazione ufficiale del partito di maggioranza nazionale e regionale, è stato un modello di gestione da imitare con zero infiltrazioni mafiose e illegalità arginata, in realtà ha mostrato non poche carenze e criticità. Nonostante questo, sono state utilizzate altrettante parole trionfali quando si è appresa la notizia che l'ex governatore dell'Emilia-Romagna, Vasco Errani, sarebbe stato nominato commissario. Forse qualcuno si è dimenticato di tutto le inchieste giudiziarie che raccontano ben altra cosa sulla ricostruzione dell'Emilia, diversa da quella osannata, anche in queste Aule, e nella quale ci sono molte zone d'ombra e molte cose che lo stesso Governo centrale e quello regionale continuano a non dire, soprattutto in tema di illegalità e inquinamento mafioso. In tal senso, negli ultimi mesi la prefettura emiliana ha bloccato 75 aziende implicate alla ricostruzione. Dietro molte di esse ci sono le 'ndrine calabresi radicate nella Regione emiliana. Come non ricordare quanto accaduto a Finale Emilia, paese vicino a San Felice sul Panaro, epicentro del sisma, in cui si è consumato un fatto di ordinaria furbizia imprenditoriale. Al centro dello scandalo la scuola media «Frassoni», da cinque milioni di euro, nuova di zecca e pronta per essere inaugurata. A distanza di quattro anni esatti, però, qualcosa nella ricostruzione non ha funzionato. Chi ha realizzato l'opera, per limare sui costi, avrebbe utilizzato il cosiddetto cemento depotenziato, materiale fragile e molto pericoloso. Così, per inquirenti e investigatori la struttura della scuola media non sarebbe sicura, tanto che ne è stato disposto il sequestro. Voglio ricordare che l'inchiesta Cubetto, dal nome che indica i campioni di calcestruzzo da sottoporre ad analisi di resistenza, è ancora in corso. Bisognerà attendere i risultati delle analisi del materiale sequestrato e poi l'incidente probatorio. coinvolte due importanti aziende, entrambe con un ruolo in Confindustria. Si tratta della Betonrossi SpA, attiva in tutta Italia e *leader* del settore, e la A&C di Mirandola, il cui proprietario, Stefano Zaccarelli, presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili di Modena, ha lasciato dopo la notizia dell'indagine a suo carico. Ma questa non è la prima ombra che si addensa sulla ricostruzione post sisma in Emilia. Anzi, è solo l'ultima di una lunga serie di anomalie. La prima, come documentato da «l'Espresso» ormai tre anni fa, è l'intromissione della 'ndrangheta nella filiera dello smaltimento delle macerie con un meccanismo molto semplice: in piena urgenza con la catena del subappalto, le strade dei paesi terremotati sono state battute dai camion dei *clan*. Hanno smaltito una quantità importante di detriti, stando a quanto scritto dagli investigatori del gruppo interforze guidato dal poliziotto Cono Incognito. Un *team*, questo, costituito ad hoc per vigilare sulle opere da realizzare nella ricostruzione e che ha lavorato sodo, prodotto decine di misure interdittive, escluso numerose aziende dalla *white list*, alcune delle quali già attive nei cantieri emiliani. Ricordo che seppure è vero che la *white list* è stata veramente un'innovazione rispetto a quello che si faceva prima, ancora non risolve, a quanto pare, tutti i problemi. Abbiamo anche il caso della Bianchini costruzioni - e mi dispiace che non vi sia il senatore Giovanardi, che di questa azienda ha parlato innumerevoli volte in quest'Assemblea *leader* nel territorio della bassa emiliana, raggiunta comunque da interdittiva antimafia quando la procura antimafia di Bologna e i carabinieri di Modena hanno scoperto la sua vicinanza alla 'ndrangheta emiliana. Così due anni dopo, i proprietari sono finiti nella maxi indagine "Aemilia" (oltre 200 indagati, ora imputati) sui *clan* calabresi emigrati nelle Province di Modena, Reggio, Parma e Piacenza. Signora

allora al punto e poi deposito l'intervento. Abbiamo sicuramente accolto favorevolmente l'aumento delle risorse, pari a un milione di euro, per l'unità che dovrà effettuare tutti i controlli, proposto dal relatore. Rimaniamo tuttavia profondamente dispiaciuti per la totale deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo, argomento

territori colpiti dal sisma rimane comunque la ricostruzione sociale delle zone delle Centro Italia; speriamo che non diventi l'ennesimo terremoto di nessuno.

ho assistito con molto sdegno alla trasmissione di Milena Gabanelli, «Report», di ieri sera, che ha dimostrato di essere tendenziosa o ignorante sulla Repubblica dell'Azerbaigian. Io sono stata scelta come osservatore parlamentare alle elezioni politiche e, successivamente, a quelle presidenziali e ho potuto constatare il modo democratico assolutamente corretto con cui si sono svolte. Forse la Gabanelli non sa che l'Azerbaigian nel 1918 è stata la prima democrazia istituita nel mondo musulmano con voto a suffragio universale, esteso anche alle donne, prima Nazione al mondo, prima della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, Paesi simbolo di uguaglianza e libertà; democrazia sospesa nel 1920 con la sua annessione all'Unione Sovietica e ripresa nel 1991 con il crollo dell'URSS. La Repubblica dell'Azerbaigian è l'unico Stato democratico musulmano al 96 per cento della popolazione ove ove le varie etnie e religioni convivono in pace, libertà e uguali diritti: uno Stato veramente laico, che dovrebbe essere d'esempio per altri Paesi musulmani. I pregiudizi espressi dalla Gabanelli sono molto lontani dalla realtà di un Paese che sta investendo molto nella formazione dei giovani e nella cultura, perseguendo i principi democratici che nel 1918 fecero nascere a Baku la prima università, la prima scuola laica per le donne, il primo teatro dell'opera. Forse le falsità dette dalla Gabanelli in trasmissione sono dovute al livore per essere stata inserita nella lista delle persone non gradite in Azerbaigian, in quanto entrata illegalmente nel Paese e nel Nagorno Karabakh, *enclave* armena il legale nel territorio dell'Azerbaigian, come riconoscono quattro risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del Consiglio d'Europa, del Parlamento europeo, dell'OSCE e della NATO, che invitano l'Armenia a ritirare le sue forze armate dai territori dell'Azerbaigian occupati, invito ripetutamente ignorato. Le trasmissioni a orologeria della Gabanelli (come quella di ieri sera sull'Azerbaigian, una repubblica con la quale l'Italia ha stretto importanti rapporti commerciali e culturali, o quella sul prosecco italiano, nel momento in cui questo vino è in testa all'esportazione, creando un grande danno economico e d'immagine ai nostri produttori, o ancora l'inchiesta sui piumini Moncler, nel momento in cui l'azienda si quotava in borsa) credo siano particolarmente inquietanti e facciano sorgere parecchi dubbi per la loro tempistica. Come diceva un noto politico italiano: a pensar male spesso ci si azzecca. E penso che la Gabanelli ci dovrebbe dare molte spiegazioni in proposito. Signora Presidente, il 22 novembre 2015 è una data che forse dice poco ai componenti di questa Assemblea e forse a molti cittadini che in questo momento ci stanno ascoltando. Questa data corrisponde al giorno nel quale il Governo ha varato il famoso decreto-legge salva banche, un provvedimento che sicuramente non ha tutelato i risparmiatori, ma anzi ha stabilito un nuovo criterio nell'affrontare le crisi bancarie, in cui si stabilisce il fatto che i cittadini non hanno più la certezza di poter vedere tutelati i propri risparmi. È stata fatta una scelta scellerata, quella di tentare di salvare quattro banche (ed è tutto da vedere se questo obiettivo verrà raggiunto), ma è stata sancita anche una certezza: i cittadini possono essere truffati impunemente e lo Stato, il Governo, non vuole e non può tutelarli. È passato un anno da quella data; quest'oggi abbiamo assistito all'ennesima protesta dei cittadini truffati, a dimostrazione che le risposte del Governo sono state assolutamente inadeguate e insufficienti. Questi cittadini non vedono ricevere il maltolto, perché non sono rientrati nelle categorie che avevano diritto alla restituzione dei propri risparmi, e anche oggi hanno manifestato nei confronti del Governo di fronte alla Banca d'Italia, per dimostrare che la realtà descritta dal Governo e descritta da Renzi non è la realtà che loro stanno vivendo sulla propria pelle. Io mi fido di più delle loro parole *(Applausi del senatore Candiani)* che dei Presidente del Consiglio che vuole raccontarci favole, ma non le può raccontare a chi è stato truffato e non è stato risarcito. Ed è tanto più intollerabile quello che sta avvenendo, a fronte di una dichiarazione di un Vice Ministro, il vice ministro Zanetti, che domenica ha dichiarato che è colpa di questo Parlamento ed è colpa della Commissione finanze se non è stata varata una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Noi abbiamo ripetutamente chiesto, in Commissione e in quest'Aula, che venisse accelerato questo obiettivo non è stato realizzato perché c'è un'inerzia evidente da parte del Partito Democratico in Commissione finanze. Noi pretendiamo chiarezza, non accettiamo più alibi, non capiamo il motivo di questo ritardo. È inaccettabile che questo avvenga, perché si ha la sensazione che qualcuno abbia qualcosa da nascondere. Se non c'è qualcosa da nascondere, si proceda immediatamente e non si permetta a un Vice Ministro di fare affermazioni offensive e che non rispecchiano la realtà dei fatti. Chi frena non siamo noi. Abbiamo sollecitato più volte, ora vogliamo delle risposte concrete.

un cancro che ha colpito il nostro Paese e sul quale dobbiamo lavorare compatti. Dobbiamo debellarlo una volta per tutte e con determinazione, ne va non solo dell'immagine ma soprattutto del futuro produttivo e ambientale dell'Italia intera. Il Veneto, purtroppo, registra un'altissima concentrazione di ecoreati: un fenomeno che è diffuso tra le medie e le grandi imprese, che spesso si liberano dei propri rifiuti al di fuori dei binari della legge. Sono episodi frequenti, quelli di inquinamento, che minano la salute dei cittadini. Proprio ieri è apparso su un quotidiano locale, «Il Mattino di Padova», la drammatica notizia di 378 nuovi casi di reati ambientali, legati che avviene in Veneto, cioè lo sversamento di Pfas, quindi sostanze chimiche pericolosissime, nelle acque. Quindi, ancora una volta, ci confrontiamo con un gravissimo episodio di inquinamento delle acque con sostanze chimiche pericolosissime. territorio a cavallo tra Vicenza, Padova e Verona. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo denunciato subito, mesi fa, questa tipologia di inquinamento che ha già contaminato l'acqua di circa 400.000 persone in tutto il Veneto

e invece l'ARPA Veneto denuncia una situazione di sotto-organico decisamente grave e inaccettabile. Le persone a disposizione dell'agenzia sono circa 200, quindi sono sufficienti a controllare solo 100-150 impianti collegati al ciclo dei rifiuti; ma in Veneto ci sono circa 1.500 impianti, quindi ci vorrebbero dieci anni per controllare una sola volta l'intera rete. È chiaro che questo è assolutamente inaccettabile. La legge che abbiamo approvato l'anno scorso è fondamentale per iniziare questo tipo di lavoro ma evidentemente non basta. Dobbiamo fare di più, dobbiamo dotare l'istituzione delle risorse necessarie a svolgere questo delicato lavoro da cui tutti i cittadini possono trarre estremi benefici. Per questo chiediamo al Governo e al Parlamento di iniziare al più presto una seria discussione su questi termini, finalizzata ovviamente ad individuare possibili soluzioni. vorrei dare lettura di una petizione presentata dagli studenti di Catania al loro rettore: «Siamo studenti per il "No" di Catania, aderiamo ad una rete nazionale che riunisce associazioni, collettivi e singoli studenti e studentesse nelle scuole e nelle università che si oppongono a questo tentativo, maldestro e pericoloso insieme, di modificare, con arroganza, 47 articoli della Costituzione. Qualche giorno fa, lei ha pubblicato una nota indirizzata a tutti i direttori di dipartimento e ai presidenti delle strutture didattiche speciali, in cui vieta espressamente la possibilità per l'ateneo di ospitare eventi sui temi oggetto del *referendum* del prossimo 4 dicembre se non in presenza di un contraddittorio con la presenza di tecnici ed esperti della materia». Ora non concluderò la lettura della petizione; il punto è che gli studenti lamentano il fatto che, secondo questa circolare, in assenza di esperti costituzionalisti, costituzionalisti, all'interno dell'università, anche laddove l'iniziativa la organizzassero le associazioni studentesche, è vietato discutere del *referendum*. Ora io mi chiedo,

luogo, se non se ne discute nelle università dove se ne deve discutere? Immagino che questa sia una iniziativa del rettore, anche se so che a Palermo c'è qualcosa di analogo.

se il Ministro abbia ha notizia che ci siano altre università che stanno dando questo tipo di impostazione e che cosa si intende fare. Dovrebbe essere scontato. A mio parere non è ammissibile che, all'interno delle università, che sono i luoghi del sapere critico per eccellenza, sia vietato discutere laddove non ci sia questa presenza magica di un esperto